Onorevoli colleghi, lo scorso 1° luglio è scomparso, all'età di 83 anni, Egidio Sterpa, membro di questa Assemblea nella XV legislatura. Nato a Vejano, in provincia di Viterbo, nel 1926, intraprese giovanissimo una brillante carriera di giornalista, entrando nella redazione del quotidiano «Il Tempo», dove fu nominato, a soli 25 anni, redattore capo. Dopo aver lavorato a «Il Giornale d'Italia», si trasferì a Milano per intraprendere la collaborazione con il «Corriere della Sera». Dopo un periodo di interruzione, nel quale accettò di dirigere il «Corriere lombardo», Egidio Sterpa tornò al quotidiano di via Solferino, in quegli anni diretto da Giovanni Spadolini. Con l'abbandono di Spadolini, motivato da un cambio di linea editoriale del quotidiano, Sterpa lasciò il Corriere e, dopo un breve rientro nella redazione romana de «Il Tempo», accettò l'offerta di Indro Montanelli di far parte di quella squadra di cronisti ed intellettuali di orientamento liberale la cui avventura giornalistica e culturale portò, nel febbraio del 1974, alla fondazione de «il Giornale». Negli stessi anni, in perfetta continuità con i contenuti ideali della sua attività giornalistica, Egidio Sterpa intraprese un più diretto impegno politico all'interno del Partito Liberale, nel quale incarnò le posizioni più moderate ed orientate ad una politica economica di segno marcatamente liberistico. Nel 1979, candidato nelle file liberali, venne eletto alla Camera dei deputati, dove fu confermato dal corpo elettorale per quattro legislature consecutive, fino al 1994. Nel corso della X legislatura fu inoltre membro autorevole del VI e del VII Governo Andreotti, in qualità di Ministro senza portafoglio con delega ai rapporti con il Parlamento. Nel gennaio del 1994 il congresso del Partito Liberale Italiano pose fine alla lunga storia di quella formazione politica, decretandone lo scioglimento, ed Egidio Sterpa, insieme ad altri colleghi di partito, prese parte al nascente movimento dì Forza Italia. Nel 2001 fu nuovamente eletto alla Camera dei deputati, ed in occasione delle successive elezioni entrò a far parte della nostra Assemblea. Nell'intenso dibattito di quella tormentata stagione parlamentare lasciò il segno di una riflessione pacata, profondamente radicata nella ragionevolezza delle argomentazioni, nel senso dello Stato e delle istituzioni e nell'orgogliosa appartenenza alla più genuina tradizione liberale, costantemente evocata nei suoi interventi all'interno di quest'Aula. Quel liberalismo, inteso come "pensiero forte" a sostegno di una certa visione del rapporto tra individuo e istituzioni e, di conseguenza, come metodo di azione per i pubblici poteri e per le forze politiche che ad esso si richiamano, costituisce il lascito più prezioso della presenza politica ed istituzionale di Egidio Sterpa. «Mai come oggi», scrisse in quel «Manifesto liberale» che costituisce il suo testamento politico, «idee e politiche liberali sono necessarie per scuotere il Paese ed allontanarlo dal rischio del declino». È allora con grande commozione e riconoscenza per un autentico maestro di quello spirito di libertà che altro non è, secondo il suo pensiero, che la condizione necessaria affinché «ciascuno sia padrone di se stesso», che invito tutti i colleghi ad osservare, in memoria di Egidio Sterpa, un minuto di silenzio e di raccoglimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord Padania, che ho l'onore di rappresentare, si associa al cordoglio espresso in quest'Aula per la scomparsa del collega senatore Egidio Sterpa, avvenuta pochi giorni fa. Egidio Sterpa è stato un giornalista attento e autorevole che, insieme ad Indro Montanelli, collaborò alla fondazione de «Il Giornale» e che svolse la nobile professione giornalistica in tanti importanti quotidiani. Anzi, si potrebbe dire a buon diritto che il giornalismo fu la sua vera passione, costellata da tanti successi professionali. Egidio Sterpa ha ricoperto nella sua lunga carriera i più alti incarichi in ambito politico ed istituzionale, sia nell'ambito della sua lunga militanza nel Partito Liberale, sia poi in Forza Italia, partito con il quale tornò in Parlamento al Senato, nella XV legislatura. Lo possiamo definire un uomo della nobile tradizione liberale, che ha vissuto in pieno la stagione della prima Repubblica ed il traumatico passaggio alla seconda Repubblica: un passaggio traumatico che lo coinvolse anche personalmente, subendo nel 1998 una condanna nell'ambito del processo Enimont. Da liberale affrontò quel processo - peraltro celebrato più sui mezzi di comunicazione che nelle aule di giustizia - con serietà e con il pieno rispetto delle istituzioni. Vogliamo ricordarlo oggi non solo per il rigore intellettuale che lo caratterizzava da buon liberale, ma anche per l'impegno e la passione politica dimostrati all'interno delle istituzioni. Un esempio di questa passione civile ci viene dalla lettura di un suo articolo, pubblicato su «il Giornale» nell'ottobre del 2007, nel quale Egidio Sterpa scriveva: «L'antipolitica dilaga e rischia di diventare un'onda che sommerge senza distinzione buono e cattivo, giusto e ingiusto». Ed aggiungeva: «Talune imputazioni ai politici sono innegabili, ma l'attacco indiscriminato al "palazzo", quasi fosse la Bastiglia, è troppo concitato e irriflessivo, nutrito in taluni casi di cupidigia smodata, manifestata con un linguaggio irresponsabile che niente ha a che fare con l'etica e la serietà». E chiudeva con queste parole: «È un assalto senza discernimento, senza razionalità, che può essere foriero della rovina totale di valori senza i quali una società e le sue istituzioni sono destinate allo sfascio». Il ricordo di Egidio Sterpa in quest'Aula ci serva per riflettere su queste sue parole così amare e così forti, ma anche così attuali e così vere. Signor Presidente, siamo qui oggi a ricordare Egidio Sterpa, giornalista e politico. Di molte persone, quando scompaiono, si dice che lasciano un grande vuoto: nel caso di Egidio Sterpa non potrebbero esservi parole più giuste. Egli lascia un vuoto che non è soltanto quello dell'uomo, quello di una vita, ma soprattutto quello della forza delle sue idee e del coraggio di crederci fino in fondo. Sterpa, che io ho conosciuto per un breve tempo, nei primi momenti della mia esperienza politica, era un giornalista e un uomo politico duro, ma disponibile. In realtà, però, è stato molto di più: è stato un vero e proprio testimone della nostra storia democratica e della tradizione liberale che ad essa ha dato molto. Nato a Vejano, in provincia di Viterbo, nel 1926, prima di impegnarsi e di entrare in politica, nel Partito Liberale, ha lavorato a lungo come giornalista: al quotidiano di Roma «Il Tempo», dove a 25 anni era già redattore capo; quindi al «Corriere della Sera», con Giovanni Spadolini. In seguito, nel 1974, ha seguito Indro Montanelli a «il Giornale». Con i liberali entrò in Parlamento per la prima volta nel 1979, schierandosi subito nell'ala più moderata,

dove è stato eletto fino alla scorsa legislatura, come ha ricordato il Presidente, e l'attività di editorialista per «il Giornale». Egidio Sterpa è il testimone della tradizione liberale italiana, un testimone del tutto originale, di un liberalismo legato all'esperienza risorgimentale e della destra storica, che ha saputo unire i valori del liberalismo anglosassone al senso altissimo della dignità dello Stato e delle istituzioni repubblicane. La sua visione liberale non era né individualista né economicista, ma era fondata sull'analisi storica e la passione morale e civile, con idee anche diverse, messe però grazie.

Il suo meridionalismo nasceva dalla conoscenza disincanta dei problemi, partecipe dei mali del Sud, mentre il suo liberismo era fondato sullo studio dei comportamenti umani e della storia, ed era per questo meno dogmatico, ma altrettanto convinto di quello di buona parte del liberalismo contemporaneo. Negli anni '70 ed '80 fu tra i pochi nella famiglia de «il Giornale» di Montanelli a tenere in vita e c'è voluto coraggio - un modo di intendere la cultura e la società che quasi tutti davano per morto. Le idee di Egidio Sterpa le conosciamo, e vi sono molti suoi libri che le tengono e le terranno ancora vive. Dell'uomo è giusto ricordare soprattutto la passione, il coraggio, la forza e l'orgoglio di non piegarsi al facile compromesso e alle mode. Come politico egli ha coniugato fermezza e pragmatismo nella sua lunga azione sempre illuminata dalla cultura e da un profondo umanesimo. La sua eredità più preziosa resta la capacità, nello scivoloso mondo della politica, di riunire, tenere assieme e valorizzare gli amici che dal suo esempio e dalla reciproca frequentazione hanno avuto tanto in questi lunghi anni. Molti di coloro che hanno seguito il suo insegnamento possono oggi andare in giro, come lui amava dire, «senza doversi togliere il cappello davanti a nessuno», come cittadini. E anche di questo dobbiamo dirgli grazie. La sua storia di grande giornalista e di liberale è quella dell'Italia.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, il 1° luglio è scomparso Egidio Sterpa: un liberale, giornalista, già Ministro e a lungo deputato e senatore della Repubblica. Un amico. Oggi commemoriamo in quest'Aula un uomo che è stato protagonista della vita pubblica della seconda metà del Novecento e di questo primo decennio del nuovo secolo. Nella sua lunga carriera da giornalista, che lo vide già molto giovane redattore capo de «Il Tempo», per poi passare al «Corriere Lombardo», al «Corriere della Sera» e a «La Notte» fino a seguire Indro Montanelli nel progetto de «il Giornale Nuovo», Sterpa mantenne sempre l'acume dell'inviato, capace di raccontare agli italiani eventi drammatici come l'affondamento dell'Andrea Doria, di cui spesso ci parlava, unito alla profondità del commentatore asciutto e a tratti spigoloso, pronto ad affermare anche le tesi più scomode, lontano da ogni cedevolezza al conformismo. È nella Milano degli anni '70 che Sterpa gettò le basi per il proprio impegno diretto in politica, facendo emergere dalle colonne de «il Giornale» un approccio liberale e pragmatico alla gestione della cosa pubblica, in un'epoca di consociativismo dominante e di illusioni collettivistiche ancora ben lungi dal tramontare. E proprio a Milano sarà eletto alla Camera dei deputati, nelle liste del Partito Liberale, nel 1979, e poi sempre rieletto sino all'ultima legislatura della cosiddetta prima Repubblica, ricoprendo incarichi di Ministro per i rapporti con il Parlamento nei Governi Andreotti VI e VII. Proprio nel difficile biennio 1992-1994 ho avuto l'occasione di conoscere personalmente e più a fondo Egidio Sterpa, e non solo come suo lettore. Ero allora il più giovane deputato della pattuglia del Partito Liberale Italiano ed ebbi l'opportunità di giovarmi dei suoi consigli e delle sue lucide analisi, nonché di scoprirne le doti e le qualità umane di cortesia e affabilità, che egli riservava solo al privato, coltivando un'immagine pubblica sobria e rigorosa. Negli anni successivi, dopo una parentesi amara, legata alle vicende giudiziarie connesse alla fine del pentapartito e alla fine della prima Repubblica, Sterpa riprese ed intensificò la peraltro mai del tutto interrotta attività di giornalista e di scrittore e aderì a Forza Italia, nelle cui liste fu eletto deputato nel 2001 e senatore nel 2006, nella convinzione di poter dare il proprio contributo liberale in un partito diverso e più ampio. Terminata anche questa esperienza parlamentare, Egidio Sterpa ha continuato, fino a pochi mesi dalla scomparsa, a far sentire la propria voce di liberale nel modo per lui più naturale: scrivendo articoli e libri uniti dal *fil rouge* dell'amore per la libertà, legato sempre e comunque ai valori della responsabilità individuale e a un profondo senso dello Stato.

Egidio Sterpa aveva seguito la propria idea di Patria, di fedeltà allo Stato risorgimentale in quella che gli era parsa l'unica scelta di campo fedele a quella certa idea dell'Italia non proprio vicina alla tradizione liberale, e meno ancora antifascista. Questo però - e mi ha fatto piacere come sia stato ricordato in quest'Aula - non ha impedito ad Egidio Sterpa di essere ricordato nella storia della nostra Repubblica come un grande parlamentare: Egidio Sterpa era uno di quei parlamentari che al Parlamento voleva bene davvero. Senatore lo fu soltanto nella XV legislatura, ed anche in Senato, dai banchi dell'opposizione (fu l'unica delle sei legislature che lo vide all'opposizione), Sterpa fece valere quella tradizione liberale in rappresentanza della quale nel 1979 era stato eletto per la prima volta alla Camera. Gli fu al fianco, nelle liste del Partito Liberale Italiano al Parlamento europeo, un grandissimo del giornalismo ancora in servizio: Enzo Bettiza.

si erano riconosciuti in quella eresia giornalistica proprio in nome dell'ortodossia del vecchio «Corriere della Sera», quello di Spadolini, che era poi lo stesso di Albertini. Alla Camera l'attività di Sterpa ebbe soprattutto due grandi punti di riferimento, uno dei quali fu il mondo della scuola. E mi ha fatto piacere che la senatrice Sbarbati abbia ricordato con tanta amicizia un giornalista che da parlamentare aveva scelto di occuparsi di scuola, di legislazione scolastica, proprio perché Egidio Sterpa sentiva che questo è il Parlamento e non la Camera delle corporazioni, e Parlamento significa che, se si è preside a direttore didattico,

Dal segretario generale Gianfranco Ciaurro ai suoi figli (di cui uno è un validissimo funzionario del Senato) c'è tutto un mondo di studi, di giovani e ormai meno giovani funzionari parlamentari che hanno avuto in Egidio Sterpa un interlocutore di studi, di articoli, di pubblicistica, di saggistica. Mi si consenta, Presidente, ancora una riflessione. al Partito Liberale, per quello che vale la testimonianza dell'ultimo Capogruppo - «capogruppetto» - dell'ultimo Gruppo liberale in Senato, la mia, le esprimo la più sentita gratitudine per aver ricordato Piero Milio ed Egidio Sterpa: un liberale del Sud e un liberale del Nord, del mondo milanese, anche se proveniva da Viterbo, da «Il Tempo» di Angiolillo e di Letta, che hanno onorato la vicenda storica e politica di quel partito e di quella tradizione. In nome di quella tradizione, Egidio Sterpa, nel 2001 e nel 2006, fece una dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo parlamentare sulla questione del Senato delle Regioni. Gli costò, ma fu bellissima: fu esemplare per sobrietà e per fedeltà a quei valori antichi del Risorgimento nazionale che sono sempre moderni. Per rispetto nei confronti dei colleghi del Gruppo alleato della Lega Nord, io la considero un modello per come si convive e si coabita in un Gruppo.

La mia amicizia con Sebastiano Sterpa e con i suoi cari mi ha conferito questa sera l'onore di esprimere, da parte del Gruppo del PdL, un sentimento di commossa

Colleghi, dovremmo ora procedere alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.

finestra"). Colleghi, in relazione all'andamento dei lavori presso la 10a Commissione,

Onorevoli colleghi,